link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Graziano Delrio, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: attuazione del nuovo codice degli appalti; problematiche relative al sistema portuale e al trasporto marittimo.

nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà. rivolgere un non formale ringraziamento alla senatrice Parente, che ha svolto un lavoro sostanziale, con il quale ha

hanno concorso, seppure con distinzioni che emergeranno nel corso dell'esame degli emendamenti, a cambiare l'originaria impostazione del provvedimento. un cambiamento che è stato suggerito dalle numerose audizioni che la Commissione ha svolto, attraverso le quali abbiamo potuto verificare quali siano le buone pratiche che, a proposito della migliore attività d'inclusione dei disabili di particolare gravità,

così posso dire, cioè un modello legislativo che chiamerei giacobino, con il quale la Camera dei deputati aveva individuato una pratica non ricorrente nell'esperienza italiana ma tipicamente anglosassone, quella del *trust*, e aveva deciso di incoraggiarla attraverso l'utilizzo dell'accantonamento effettuato in seno alla legge di stabilità. La scelta opposta, che la Commissione ha compiuto, è quella di una legge che chiamerei capacitatrice della vitalità della nostra società; una legge con la quale, cioè, prenderemmo atto, ove confermata dal voto dell'Assemblea, delle attitudini che nelle nostre comunità si sono manifestate, soprattutto con iniziative di carattere solidale, dando ad esse quell'ulteriore supporto affinché si diffondano quanto più. È una scelta ben diversa di legiferare, che si rifà all'idea di uno Stato che non pretende di sostituirsi alla società, che riconosce le attività sussidiarie e attraverso di esse realizza quel progetto di deistituzionalizzazione delle risposte ai bisogni di inclusione e di autosufficienza dei gravi disabili. Questo modo di legiferare è, appunto, l'esatto opposto di quello che ho definito giacobino, perché con esso lo Stato tende a sostituirsi alla società o pensa di avere di avere in sé la capacità di discernere la virtù e pensa di doverla imporre alla società. Sono due cose diverse.

ampio menù di opportunità che liberamente la società potrà scegliere, tutte ugualmente sostenute attraverso una fiscalità amichevole e altre forme di sostengo. La seconda considerazione che desidero fare è riferita a una norma di principio che ho io stesso proposto che è stata corretta dal Governo. Ho accettato la correzione, anche se devo ritenere che la norma da me proposta non sia stata ben compresa dal Governo nel momento in cui ne ha chiesto quella correzione. Ho proposto il richiamo a quei principi dell'ordinamento che sono variamente codificati e che troviamo in particolare nella legge sul federalismo fiscale, secondo i quali in ogni contesto territoriale la dimensione sanitaria si dovrebbe integrare quanto più con una dimensione sociosanitaria o sociosanitaria assistenziale, affinché la presa in carico della persona, cui sempre facciamo riferimento, conduca alle risposte più appropriate ai bisogni che la persona manifesta, a partire innanzitutto da quel dovere di prevenzione del formarsi di uno stato di bisogno. Ebbene, nella legge sul federalismo fiscale e nei provvedimenti che ne seguirono noi individuammo la ideale proporzione tra i macrolivelli di assistenza. Mi riferisco innanzitutto alla prevenzione, che identificammo nel 5 per cento della complessiva spesa sociosanitaria assistenziale di un territorio,

che sono così consoni ed appropriati per i bisogni di cui ci occupiamo in questo provvedimento. Infatti, potremo dare valore alle modeste risorse che qui stanziamo che qui stanziamo per i gravi disabili se le collocheremo nell'ambito di una organizzazione della spesa sociosanitaria assistenziale quanto più efficiente e corrispondente a quei macrolivelli di assistenza. Il Governo non si deve preoccupare del richiamo a quei principi, come ha fatto chiedendomi di aggiungere soprattutto l'invarianza della spesa, in realtà, il richiamo a quei principi significa riduzione della spesa per spedalizzazione inappropriata, chiusura di plessi ospedalieri pericolosi perché al di sotto delle soglie minime di efficienza e potenziamento corrispondente della spesa per servizi territoriali che, come dicono quei macrolivelli di assistenza che il Presidente conosce molto bene, avendo concorso in prima persona alla legge sul federalismo fiscale, vogliono che il 51 per cento della

determina inappropriatezza di ricoveri rispetto a persone che devono trovare invece strumenti di autosufficienza e di inclusione in altre prestazioni e in altre opportunità, come quelle che qui vogliamo sostenere e diffondere.

e chiede che ci sia uno spostamento di spesa dalla dimensione ospedaliera alla dimensione del territorio, così come nelle buone pratiche italiane possiamo riscontrare. Sono orgoglioso di venire da un territorio nel quale l'azienda integrata di servizi sanitari e sociosanitari, da circa dieci anni e forse più, è in avanzo di gestione proprio perché realizza alti livelli di appropriatezza ed offre risposte più appropriate

in certa misura, quasi occasionali, diventano strutturali, perché si inseriscono nel giusto contesto. Non sono i 90 milioni di cui stiamo discutendo che cambieranno la condizione dei disabili gravi, ma possono essere un utile volano se collocati nell'idoneo contesto istituzionale. Di questo fa parte anche l'integrazione tra la spesa sociosanitaria dei Comuni e l'attività delle aziende sociosanitarie integrate dei territori. Nella nostra esperienza veneta, i Comuni conferiscono la loro spesa alle aziende integrate che la gestiscono con contabilità separata sotto l'indirizzo dei sindaci, ma sostanzialmente garantiscono piena sinergia tra la dimensione sanitaria e quella sociosanitaria. Con queste caratteristiche mi auguro che il provvedimento possa raggiungere un ampio livello di consenso, ben superiore a quello dei confini della maggioranza, corrispondendo, spero, il voto dell'Assemblea al dialogo che costruttivamente si è svolto in Commissione e per il quale rinnovo il mio ringraziamento a tutti i Gruppi, davvero nessuno escluso, perché tutti hanno concorso a cambiare l'originario testo di legge. Presidente, ci troviamo di fronte un provvedimento che apparentemente ha un nome che evoca delle sensazioni di solidarietà («Dopo di noi»). siccome è una proposta che deriva da una forza politica in cui non ho assolutamente fiducia, bisogna

Questa norma recita: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione». Bene, andiamoli a vedere. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale». depurato l'articolo 2 della nostra Carta costituzionale delle parole che, nel contesto riferito a questo provvedimento legislativo, non non hanno pertinenza, in modo tale che diventi più semplice la lettura, a fronte dell'ispirazione che questa norma richiama. si cita l'articolo 3 che, per antonomasia, è l'articolo sull'uguaglianza: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione (...) di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

rimanda al coinvolgimento dei soggetti interessati ma nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Parole saggissime dei nostri Padri costituenti. Prosegue provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato». Difatti, l'articolo si cita in questo provvedimento e quindi questi 90 milioni dovrebbero servire anche a fare questo. andiamo avanti, perché poi riprenderemo il discorso dei 90 milioni.

prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari (...) e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà». Questo è un inciso fondamentale non inserito nel provvedimento in esame. Magari qualcuno potrebbe dire dire che non ce n'era bisogno, perché non si tratta assolutamente di provvedimenti che vanno a incidere sull'eredità. Ah! «Dopo di noi», che bel nome! Ovviamente, la prima cosa che viene in mente è: fantastico, facciamolo! Bellissimo, introduciamolo! Ora, però, capisco cosa c'è dietro. Perché avete bocciato questi emendamenti che cercavano di introdurre tale principio nel disegno di legge? Perché in un disegno di legge, che tra le buone norme che potrebbero dare sollievo - se attuate rapidamente, ma poi vedremo, che non lo saranno saranno - prevede proprio norme che gestiscono l'eredità non inserite tra i principi ispiratori anche quello che assicuri l'eredità e gli affari finanziari e quello che precisa che le norme devono assicurare che le persone con disabilità

privazione dell'eredità delle persone con disabilità grave, trasformando così il problema delle persone in una nuova forma di mercato. Signor Presidente, soltanto

quella dell'assistenza ai disabili privi del sostegno familiare era una lacuna che andava colmata già da molto tempo. Il disegno di legge, approvato in prima lettura alla Camera con il voto favorevole di tutti gli schieramenti, tranne il Movimento 5 Stelle, è volto a introdurre nel nostro ordinamento l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave che perdono il sostegno familiare a causa dell'invecchiamento o della morte dei genitori.

di un problema serio, trascurato per decenni, che vede coinvolte almeno 580.000 persone affette da disabilità grave. Tuttavia, se il punto di analisi si estende ad altre forme di disabilità, si vedono numeri elevatissimi,

istituire un fondo per l'assistenza e prevedere regimi fiscali agevolati per la tutela del patrimonio destinato all'assistenza del disabile. In particolare, attraverso l'istituzione del Fondo finanziato con 90 milioni di euro per il 2016 (è già stato detto qualcosa in proposito), 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro a partire dal 2018, si dovrebbe dare la possibilità al disabile di continuare a vivere nella propria abitazione o in case famiglia, anche dopo la perdita dei genitori. Inoltre, è previsto che non sia sottoposto a tassazione tutto ciò che i genitori destinano ai propri figli sotto forma di coperture assicurative, Ebbene, è proprio sulle modalità di finanziamento e utilizzo del suddetto Fondo che forse si dovrebbe essere un po' più chiari. prevede, inoltre, iniziative volte ad agevolare la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative con le indicazioni specifiche di progetti che abbiano come obiettivo prioritario la vita indipendente delle persone disabili, integrando le risorse a cui hanno diritto. Oltretutto, per i disabili gravi privi di sostegno familiare sono previsti progetti mirati alla creazione di famiglie comunità e di case famiglia in cui inserire le persone che lo desiderano. È proprio sulla possibilità di acquisto di nuove case da parte degli enti su cui si possono esprimere altre perplessità. Il disegno di legge presenta quindi alcuni aspetti su cui bisogna vigilare, tenendo alta l'attenzione sull'effettiva implementazione. Infatti, si legge nel testo del provvedimento che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. necessario un intervento tempestivo del Governo, affinché tutte le misure predisposte nel testo legislativo in esame possano essere applicate nell'immediato. Bisogna vigilare sulle risorse messe a disposizione dei disabili affinché siano effettivamente loro destinate, evitando che si disperdano in imbuti burocratici e rivoli farraginosi. A questo riguardo, accogliamo con favore la disposizione contenuta nell'articolo 8, in cui viene stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve relazionare con cadenza annuale sullo stato di attuazione delle misure previste e dell'effettivo andamento delle risorse destinate ai disabili.

politiche e richiesta dall'opinione pubblica, ma non va dimenticato che i genitori che si prendono cura dei figli disabili hanno bisogno di assistenza durante la loro vita, che dedicano, con assoluta devozione e abnegazione, alla cura del familiare disabile. Pertanto, auspichiamo che il Parlamento, una volta approvato il disegno di legge sul "dopo di noi", prenda in esame i disegni di legge sul *caregiver* familiare e avvii l'ordinario *iter* legislativo. Bisogna rendersi conto che nel nostro Paese ci sono 9 milioni di persone che si dedicano all'assistenza di un familiare non autosufficiente. Eppure, l'assenza di riconoscimento della figura del *caregiver* familiare e della possibilità di anticipare il pensionamento per dedicarsi alla cura

la Camera aveva approvato il disegno di legge che consentiva ai *caregiver* familiari di andare in pensione una volta maturato trent'anni di contributi e almeno diciotto anni di assistenza continuativa ad un disabile. È ora di riprendere queste iniziative e portarle a termine. In conclusione, siamo lieti di accogliere questo provvedimento. Auspico che ci sia una volontà comune nel dare, al più presto, tutto il supporto necessario, in termini di assistenza, anche ai familiari che dedicano un'intera vita all'accudire i parenti disabili. Il nostro, doveroso, rispetto nei confronti di chi ha bisogno di aiuto non deve rimanere confinato nelle solite parole di solidarietà e vicinanza, ma deve tradursi nell'impegno concreto di provvedere a forme di assistenza, sostanziali e congrue, sia per i disabili che per i familiari. Mi auguro che gli intendimenti del legislatore non siano frustrati da formulazioni poco chiare o da successive farraginosità burocratiche che rendano questo provvedimento poco trasparente. È per questo motivo che ho presentato alcuni emendamenti, che spero vengano accolti. *(Applausi

innanzi tutto vorrei ringraziare la relatrice che mi siede a fianco per il lavoro svolto in Commissione, dove trasversalmente abbiamo cercato davvero in tutti i modi di trovare sempre la sintesi

ci hanno permesso, oltre all'ascolto, anche un confronto proficuo, e non è stato facile perché in alcuni casi davvero ci siamo emozionati e commossi. Oggi è davvero una giornata importante, come è stato ricordato da molti colleghe e colleghi, per molte persone che nel nostro Paese sono in grave difficoltà e *deficit*. è anche per tutti noi, non soltanto per i disabili e per le loro famiglie. È una giornata importante per tutti coloro che vivono e convivono con una disabilità grave, che alla fatica quotidiana, aggiungono un'angoscia, cosa avverrà negli anni successivi, quando coloro che accudiscono queste persone non ci saranno più. Ecco, quindi, che è utile in questa sede analizzare le ragioni delle scelte fatte, che sono all'origine di un provvedimento anni fa dalle famiglie, arriva dal basso, in particolare da alcune grandi associazioni di familiari di persone con disabilità cognitiva e da tante piccole esperienze di "dopo di noi" diffuse su tutto il territorio nazionale, tra le quali anche il mio territorio di provenienza, il Piemonte, dove sono già operative alcune esperienze in questo senso. Ad esempio,

La richiesta dei soggetti citati fu raccolta dall'onorevole Turco nella precedente legislatura, ma il problema grandissimo che non riuscirono a superare fu, come succede spesso, di risorse. Si prevedeva, infatti, in una prima fase un miliardo di risorse e la platea era molto più allargata. In questa legislatura si è, quindi, ripreso l'*iter* interrotto (era una promessa fatta), si sono ridotte le azioni e anche la platea

prima volta in questa legislatura che ci sia prima una posta di risorse e dopo l'approvazione di un provvedimento. Si tratta, quindi, di una conquista, ma, proprio per la quantità dello stanziamento (90 milioni), non si può ancora parlare di una riforma del sistema. Si è, però, cercato di mantenere il nuovo cambio di prospettiva e di continuare in una direzione intrapresa. È quindi un percorso, quello che si sta facendo. L'articolo 2 mantiene infatti l'obiettivo

con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento» è stato operato proprio grazie alla segnalazione del mondo associativo. Non bisogna confondere la platea del provvedimento con i 2,5 milioni di persone attualmente non autosufficienti e anziani. La disabilità grave, statisticamente, è soprattutto cognitiva o psichica e la stessa capacità di autodeterminarsi è limitata e spesso interviene l'amministratore di sostegno, il cui ruolo di collegamento con il *trustee* è stato previsto nel provvedimento arrivato in Assemblea dalla Camera

disposizione sta davvero finendo. Certamente si dovrebbero approfondire di più la condizione delle famiglie, che sono sempre più piccole, fragili e monogenitoriali, e l'opportunità di un'offerta plurima di servizi, comprensiva

in esame propone un percorso verso il massimo di autonomia raggiungibile a seconda del livello di disabilità e quindi completa e non sostituisce la legge sulla vita indipendente già citata, n. 162 del 1998. citare anche che esso tiene conto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che recita, alla lettera *a)*: «Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove

intende promuovere la vita indipendente, che non è in contrasto con la scelta di vivere in piccoli gruppi. Potenziare questa opportunità non significa infatti segregare nessuno, se questo è l'ambiente che corrisponde al meglio, al progetto di vita delle persone che lo scelgono. citare ancora il mantenimento dei 400 milioni di euro nella legge di stabilità per il Fondo nazionale la non autosufficienza, di cui una parte è dedicata proprio al sostegno dei programmi di vita indipendente. Ricordiamo che abbiamo anche ottenuto 5 milioni di euro aggiuntivi, proprio con la legge n. 162 del 1998. di una legge molto pratica, che risponde a richieste specifiche e a bisogni concreti, ma che non si pone in una logica di riforma complessiva di tutto il sistema, anche se è orientata verso un sistema sociale rispettoso delle persone - voglio sottolineare questo

dice: «Sono molto felice di vedere che il progetto in cui con molti di voi ho creduto in questi anni sta prendendo vita, perché alcuni ragazzi hanno iniziato a vivere l'esperienza di vita indipendente quattro giorni la settimana. Non solo. Come certamente avrete avuto modo di vedere alla TV o sui giornali il nostro Governo sta approvando una legge che va proprio nella direzione che noi abbiamo avviato. Di questo ringrazio il Signore e auguro a tutti i genitori di trovare il coraggio di guardare ai loro figli come adulti, scoprendo che in ognuno di loro Dio ha messo delle cose meravigliose che noi dobbiamo imparare a vedere e a far emergere*».

dal dibattito in quest'Assemblea, molto interessante e proficuo, è emerso che anche chi ha avuto toni e accenti più critici non ha potuto non sottolineare la bontà di questo disegno potrei citare i colleghi che l'hanno fatto). Infatti, è difficile criticare un disegno di legge che per la prima volta nella storia legislativa italiana parla del destino delle persone con disabilità. Da domani, da quando sarà approvata la legge, (e non è cosa da poco) le famiglie delle persone con disabilità, o chi le rappresenta e ne tutela gli interessi, potranno andare presso l'ente locale o il Comune

nulla, ma si integra e si aggiorna. Come? Anche con un fortissimo sistema valoriale, nonché con l'aggiornamento e l'adeguamento della nostra legislazione agli *standard* europei e internazionali. Qual è il valore profondo vi sia riferimento a tutti gli articoli della Convenzione

il fondo servirà anche a questo. L'ultima questione è quella che ha ricevuto maggiori critiche (penso al Movimento 5 Stelle e alla senatrice Serra). Abbiamo modificato sostanzialmente l'articolo 6 che riguarda la questione dei *trust*. Stiamo parlando di segregazione patrimoniale; vuol dire

il *trust* non è contemplato dal nostro codice civile e ha un impianto di tipo anglosassone. La senatrice, ad esempio, faceva riferimento al contratto di affidamento fiduciario, previsto possa essere gestito anche da società fiduciarie e da ONLUS con specifico obiettivo della beneficenza.

non ce l'ha. Questa è stata la principale modifica che abbiamo apportato al Senato e questo ci sentiamo di aver fatto. Abbiamo legiferato e modificato il testo in Commissione. Anch'io ringrazio tutte

Signor Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a concludere è frutto di un lungo lavoro, condiviso da tanti Gruppi, al quale anche il Governo ha dato il proprio fattivo apporto. Ciò nella consapevolezza della necessità di prevedere disposizioni a tutela della persona con disabilità grave, anche nel momento in cui venga meno il sostegno familiare, in un percorso ideale la cui tappa finale è il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia della persona. Le disposizioni recate dal disegno di legge, vorrei ribadirlo, hanno come finalità quella di garantire il superiore interesse delle persone con disabilità grave, come recita appunto l'articolo 1. Allo stesso tempo si fornisce una risposta, da tanto attesa, a quelle famiglie che vivono oggi l'inquietudine, l'angoscia, la preoccupazione e lo sgomento nell'immaginare la vita dei loro cari in un futuro senza la loro presenza. È questa l'essenza del "dopo di noi" Oggi, con l'approvazione di questa legge, stiamo facendo qualcosa di estremamente importante. Questo provvedimento influirà positivamente sulla qualità della vita delle persone gravemente disabili e dei loro familiari. Per la prima volta si danno risposte concrete a quelle famiglie, in particolar modo a quei genitori, spesso anche anziani, che si sono presi cura del proprio figlio o della propria figlia, gravemente disabile e che quotidianamente vivono con l'angoscia e il tormento, ponendosi l'interrogativo di chi si occuperà dei loro familiari disabili quando loro non ci saranno più o quando non saranno più in grado di assisterli. È un provvedimento centrato sulla persona. Io penso che tutti noi, abbiamo persone vicine, amici, parenti, conoscenti (anche chi vi parla) che vivono questa difficile realtà. Credo che le vere barriere quotidiane che un disabile incontra non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle culturali ed oggi con questo provvedimento possiamo dire di aver fatto anche un balzo culturale sì, io credo che sia soprattutto un gran balzo culturale - che permetterà di garantire sia una qualità della vita sia una vita futura alle persone con disabilità. Come ho detto, ci sono leggi che segnano anche una svolta culturale ed è il caso di questa legge. Abbiamo istituito un fondo di 90 milioni per quest'anno affinché tutti i soggetti interessati possano assicurare dei percorsi personalizzati per i disabili gravi dopo la morte dei genitori; progetti di vita personalizzati (mi rendo conto che se il fondo fosse più cospicuo sarebbe meglio) decisi dai genitori, da fratelli e sorelle, e dai protagonisti stessi, quando il tipo di disabilità glielo consente. Finalmente si riconosce il diritto che le famiglie del disabile hanno atteso da tempo: decidere il luogo e il modo in cui esso vivrà. La condizione di disabilità non riguarda solo le persone che che ne sono colpite e le loro famiglie, ma anche la comunità e le istituzioni, che devono operare in stretta collaborazione, in rete nei diversi livelli di responsabilità.

si possa dare una risposta per le progettazioni sperimentali che si realizzano esclusivamente durante la vita in famiglia delle persone con disabilità. Al finanziamento di questi programmi e di questi interventi possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, nonché i soggetti di diritto privato. Con questa legge diamo alle famiglie e alle persone con disabilità la possibilità di avere un futuro migliore e più sereno. Abbiamo messo a disposizione risorse - forse ce ne vorranno di più, me ne rendo conto - e strumenti che non vogliono imporre comunque un percorso *standard*, ma diversi percorsi. Per ciò che concerne le disposizioni finanziarie, l'articolo 9 del provvedimento prevede 90 milioni per il 2016 (già previsti nella legge di stabilità), 38 milioni per il 2017 e 56 milioni a decorrere dal 2018.

Personalmente, è una vita che cerco di occuparmi di disabili. Per me è un passo avanti ed è un passo avanti per le nostre famiglie. So che molti di voi hanno dei familiari

di una parte dell'emendamento: «Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche».

tempo, ci parrebbe giusto che questa vostra creatura fosse accettata anche in questa sede; sarebbe quindi schizofrenico non accogliere il suggerimento. Con l'emendamento 1.19 chiederemmo di spingerci

ma che contiene la solita furbata consistente nel far entrare dalla finestra uno strumento utile solo a chi manovra soldi, grandi soldi, ma che non ha nessuna finalità né umana, né filantropica, né pubblica. *(Applausi

Noi sappiamo che il provvedimento in esame è diretta alla protezione dell'interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare o perché i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

che cerchiamo di risolvere il problema di poche decine di persone in Italia che hanno avuto la sfortuna, circa cinquant'anni fa, di nascere focomelici per la questione del talidomide. soggetti, all'interno di un periodo predeterminato, hanno avuto l'accompagnamento: me ne interessai a suo tempo quando ero al Governo.

ma gli anni passano e questa discriminazione nei loro confronti diventa sempre più odiosa. Stiamo parlando di qualche milione di euro, non di miliardi di euro. non questo provvedimento perché emendamenti al riguardo non ne sono stati presentati, ma un provvedimento gemello in Commissione sanità. Il Governo per cortesia

Cerchiamo insieme di dare una risposta a questo problema.

parole, sia a rischio l'eredità delle persone con disabilità grave. Evitate allora questo mio mal pensiero perché, a volte, a pensare male si fa peccato ma molto spesso

chiedono a ciascuno Stato di proteggere, assicurare l'eredità delle persone con disabilità e di normare affinché ci sia una completa protezione.

le parole: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno». Questo emendamento ci appare opportuno in quanto in esso facciamo un richiamo all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si occupa di diritti dei bambini in generale e, quindi, anche di bambini con disabilità e della loro piena inclusione, da garantire sin dalla prima fase della vita. Occorre anche, come fatto con l'emendamento proposto, focalizzare meglio l'attenzione sulla necessità di attivare percorsi di autonomia sin dalla minore età, preparando il periodo dell'età adulta e quello successivo del cosiddetto "dopo di noi", ossia da adulti senza più il sostegno familiare, attraverso un graduale e continuo percorso di crescita, declinandone il progetto individuale che ciascuna persona con disabilità,

che appare per noi decisamente limitativo, a fronte delle reali esigenze delle persone disabili nel nostro Paese. Infatti, le condizioni di debolezza, di fragilità e di necessità in cui può trovarsi una persona disabile non possono essere ricondotte *tout court* esclusivamente ai casi di disabilità grave. Tale scelta legislativa appare appare quindi per noi miope e meritevole di un intervento di più ampio respiro, anche perché non esiste una definizione precisa

provvedimento è composto da tre commi: i primi due ribadiscono cose già previste da altre leggi e l'unica novità è quanto previsto dal comma 3, ovvero l'istituzione del *trust,* che permetterà alle famiglie di lasciare i loro patrimoni a fondazioni private che gestiscono istituti.

parere contrario su tutti gli emendamenti

vorrei spiegare al meglio cosa intendiamo fare con questo emendamento, sempre per far capire la gravità della scelta di concentrarsi solo ed esclusivamente su una piccola platea di aventi diritto. Rimarchiamo ancora una volta che i LEP sono stati stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Il fatto di non voler mettere in pratica la Costituzione rende questo provvedimento veramente piccolo: un'occasione mancata di fare la Storia. concentrati su un piccolo problema, nel momento in cui avete avuto l'occasione di sistematizzare questioni rimaste in sospeso, in particolare per quanto dice la Costituzione. Questo, a nostro avviso, è molto grave e con l'emendamento in titolo vi diamo l'opportunità di rimediare alle mancanze strutturali del disegno di legge.

perché il Movimento 5 Stelle ritiene che, prima di andare a creare nuovi istituti giuridici di diritto privato, per favorire magari una platea di 1.500 disabili, a fronte di una platea allargata di 300.000 persone,

a nostro avviso, non possono esserci limiti economici per i livelli essenziali

ai fini della piena ed effettiva realizzazione del progetto etico e normativo contenuto nel presente disegno di legge, è da considerarsi opportuno programmare in modo sostanziale azioni e scelte tecniche che realizzino pienamente la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità per le persone con disabilità prive di sostegno familiare, che risiedano in soluzioni abitative che non garantiscano garantiscano condizioni di libertà e di dignità tali da soddisfare la piena realizzazione della persona umana*.

L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinata alla sussistenza dei requisiti che andrete a individuare in un secondo momento. il nostro emendamento 3.6 chiediamo la soppressione di tale comma, per evitare di trovarci, al solito, con un Governo che ha le mani talmente libere da poter fare, vincolare e destinare in modo troppo discrezionale.

di denari che spesso nel nostro Paese si inabissano in rivoli torbidi e deviati. Ci sembra il minimo che dobbiamo ai cittadini che necessitino di cure e attenzioni. Chiediamo, quindi, la certezza del percorso del Fondo, tramite verifiche di trasparenza e tracciabilità.

questa normativa «è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1». Già abbiamo visto il trucchetto che

il comma 2. Ne chiediamo la soppressione, perché, come al solito, al Governo e alla maggioranza si lasciano le mani libere. Si lasciano le mani troppo libere per poter far destinare, vincolare e definire chi potrà accedere alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo, con subordinata la sussistenza di requisiti da individuare con l'ennesimo decreto. Per cui ci piace tanto delegare e ci piace così tanto poi non dire che cosa andremo a delegare, ovvero quali sono questi requisiti. Faccio un esempio: l'accreditamento delle residenze sanitarie assistite. Anche in Toscana, un accreditamento è come un diamante, è per sempre.

questo praticamente non è più revocabile, perché non esiste una legge regionale e nazionale che prevede la revoca dell'accreditamento. Quindi, dopo questi pasticci che sono stati fatti negli ultimi dieci anni, a fronte di tutti gli scandali che quotidianamente abbiamo denunciato e che avvengono spesso e specialmente al Sud, non sarebbe tollerabile sentirsi ancora dire: sì, ma l'accreditamento non si può revocare. Ecco, non vorremmo che venisse fatto l'ennesimo pasticcio nell'assegnazione dei soldi a questo Fondo. Per questo chiediamo di sopprimere il comma 2.

con il fondo per la non autosufficienza c'è stato sempre il problema della tracciabilità dei fondi. Al Sud e non solo, a volte, per mancati trasferimenti o per ritardi, i soldi si inabissano chissà dove. E allora, per dare un miglior per dare un miglior contributo, stiamo semplicemente proponendo di inserire la tracciabilità di questo nuovo Fondo, anche se siamo contrari al fondo

Signor Presidente, noi capiamo che, quando in questo Parlamento viene riportato in un disegno di legge un aumento di risorse, questo è considerato da tutti

nazionale per la non autosufficienza. Tutti noi ricordiamo il famoso Libro bianco di Sacconi - che se non sbaglio è colui con cui state facendo questa legge - e i tagli tremendi che fecero, lui e Tremonti, al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche

delega che affidiamo al Governo. Non sono infatti assolutamente chiari i processi di deistituzionalizzazione per il rientro e il mantenimento dei soggetti anche presso il proprio domicilio o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensioni ristrette che possono riprodurre l'ambiente

4.15 vorrei ribadire il concetto che avevo espresso prima. Tra le finalità del Fondo c'è quella di attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione.

lettera *b)*, leggo: «realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza».

previa autorizzazione del disabile stesso, qualora goda delle proprie capacità mentali, o di un tutore che se ne prende cura. Pertanto, se c'è una mamma con un disabile che si rompe una gamba,

«abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate a un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile».

è un inizio, una possibilità. Una delle cose che non riusciremo ad avere con questo disegno di legge sono proprio le attiviamoci in maniera positiva con questo circolo virtuoso. Non sarà per l'anno prossimo, perché sappiamo che i finanziamenti arrivano negli anni successivi, quindi aspettiamo; però iniziamo,

percorsi di supporto alla domiciliarità, favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, quindi per dare ordini di priorità precisi. Un rafforzamento che troviamo anche nell'emendamento 4.19, nel quale si specifica chiaramente che i programmi di intervento che andranno a favorire i percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità saranno presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o nella quale ha stabilmente il domicilio. Tutto ciò è ancora più marcato nell'emendamento 4.22, là dove si tende a dare opportunità nelle condizioni abitative

vorrei cercare di attirare l'attenzione dell'Assemblea perché tra le finalità del Fondo, come prevede appunto l'articolo 4, c'è la possibilità di acquistare immobili. Dal momento che tutti i Comuni di appartenenza possiedono immobili (basti pensare a quello che è successo con il Comune di Roma), penso che l'acquisto il Comune di Roma), penso che l'acquisto di immobili per favorire percorsi di deistituzionalizzazione sia da prendere in considerazione solo quando il Comune non abbia disponibilità di immobili abitativi da mettere a disposizione.

seguente proposta di riformulazione: «*Sostituire la lettera* b*) con la seguente*: "*b)* realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare

Visto che stiamo parlando di deistituzionalizzazione, è opportuno andare a inserire in maniera particolareggiata, per evitare pensieri cattivi, quanto segue: «Preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità». Va bene, quindi, attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire i percorsi di deistituzionalizzazione, ma segnaliamo una preferenza, che è quella dell'abitazione di origine della persona con disabilità.

so che per molti di voi ho già portato a casa troppo, ma la sostituzione di *co-housing* con la dizione «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi destinati a un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile» non mi sembra così

volte alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto di locazione, di ristrutturazione, eccetera.

regioni assicurano la vigilanza costante delle strutture atte alla gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi

il mio ordine del giorno chiede al Governo che vi siano interventi, anche normativi, qualora il disabile sia supportato dalle famiglie

Presidente, intervengo per ribadire i concetti che ha già espresso la senatrice Bencini. Il tema posto dall'emendamento 4.0.4 è proprio questo: nella parte riservata allo Stato,

che andrebbero, secondo le stime dell'ISTAT, alle persone con disabilità, per affrontare addirittura una ristrutturazione abitativa

la norma è stata inserita all'articolo 9, contrario su tutti gli emendamenti

il *trust,* che avete sviscerato con più amore e dedizione degli altri. Nel bel mezzo di un disegno di legge che verrà ricordato con la bellissima espressione del "dopo di noi", ci troviamo infilato dentro un nuovo istituto giuridico che nemmeno era stato concepito nella mente del proponente iniziale del disegno di legge.

vi dà la possibilità di evitare l'ennesima forzatura legislativa alla quale avete ormai abituato quest'Assemblea, con l'abrogazione totale dell'articolo 6 e la conseguente rimessa al mittente della bravata, o meglio della furbata da questo strumento individuale che consente di spossessarsi, con agevolazioni fiscali, di patrimoni propri a vantaggio di un beneficio futuro. Se la traduzione della parola «*trust*» è fiducia, ci chiediamo quale fiducia potranno avere gli italiani nei confronti di tutte queste forzature che, a conti fatti, soddisferebbero solo 1.430 persone Per arginare questa emorragia abbiamo presentato emendamenti sostitutivi,

a sostegno dei disabili, per questo disegno di legge "dopo di noi", il *trust* con esenzioni e benefici fiscali e patrimoniali, l'emendamento 6.322 propone di varare, con un decreto del Ministro dell'economia, disposizioni per evitare il verificarsi che un *trust* venga costituito con la preminente finalità di beneficiare di esenzioni fiscali e patrimoniali

contrario su tutti gli emendamenti

Presidente, non vorrei essere eccessivamente pedante, ma, siccome i colleghi del Movimento 5 Stelle ogni volta che qualcuno di noi si permette di votare per il collega, che magari è a due metri, obiettano e ne hanno ragione, è inaccettabile che il voto sia dichiarato da un soggetto, che è pure Capogruppo, perché il voto è personale. Come la tessera è personale, anche il voto è personale. Quelli che sbagliano dicano che hanno sbagliato.

Signor Presidente, siamo tutti un po' stanchi e i facili applausi che il senatore Buemi strappa in queste occasioni mi sembrano inopportuni. Lo inviterei ad estrarre la pallina che ha all'interno della sua buchetta e all'interno delle buchette della maggioranza.

di poc'anzi e chiedo che tutti quanti ci alziamo in modo da dichiarare il voto e lo faremo per ogni votazione, così il senatore Buemi starà qualche annetto in più incollato alla sua poltrona. Però schiacci il bottone.

che non hanno avuto e continuano a non avere risposta. E allora, purtroppo, ritorno ancora alla solita litania, signor Presidente, di un Governo che non

perché si ispirano a un ruolo positivo e utile dell'interlocuzione tra Parlamento e Governo, che reputo molto importante perché valorizza la funzione parlamentare anche in relazione alle rappresentanze territoriali», poi ha aggiunto: «Ricordo, per esempio, che alla Camera dei deputati la seduta del venerdì mattina è dedicata agli atti di sindacato ispettivo Ovviamente, come Governo non mi posso permettere di intromettermi nell'organizzazione dei lavori. Quello che posso dirvi è che, qualora l'organizzazione cambiasse, siamo assolutamente disponibili a corrispondere alle maggiori e puntuali necessità poste dai colleghi con le mozioni».

«Eh già, io sono ancora qua». Sono ancora qua per intervenire continuamente, finché il Governo non si assumerà l'impegno nei confronti dei parlamentari e dei cittadini. Per cortesia, Governo, rispondi a queste interrogazioni!

come noto il 5 giugno prossimo si svolgeranno in oltre 1.300 Comuni del nostro Paese importanti elezioni amministrative. In Sardegna andranno al rinnovo 101 amministrazioni Quando sono indette elezioni, ancorché locali, lo Stato ha il dovere di assicurare a tutti gli elettori (che si tratti sia di residenti nel territorio nazionale, nazionale, sia di residenti all'estero) l'esercizio del diritto al voto, così come garantito dalla nostra Costituzione. I trasporti tra la Sardegna e quello che noi sardi chiamiamo, con un'espressione generica, il continente sono un problema quotidiano per tutti coloro che vogliono lasciare o arrivare nell'isola. Il Governo, tra l'altro, si è impegnato anche recentemente con consistenti risorse per assicurare la continuità territoriale per tutti i sardi. Eppure, nelle prossime settimane è già prevista la pressoché impossibilità di prenotare un biglietto aereo per la nostra Regione, anche per quello che gli operatori turistici chiamano ponte vacanziero. Ovviamente questa è una buona notizia, perché significa che molti turisti hanno scelto di passare dei giorni di vacanza in Sardegna. se nelle prossime ore non ci sarà un intervento non solo della Regione (tra l'altro ampiamente impegnata), ma anche del Governo nazionale, per superare questa situazione, per migliaia di emigrati sardi, cittadini italiani che hanno mantenuto un rapporto stretto con le proprie radici e la propria Regione, risulterà impossibile esercitare quel diritto al voto che molti dei nostri corregionali ritengono ancora un loro diritto civico. Sono proprio gli emigrati che, in queste ore, attraverso le loro associazioni, ci stanno chiedendo di intervenire in fretta con le principali compagnie aree che assicurano le rotte per la Sardegna. Mi auguro e confido nel fatto che nei prossimi giorni il Governo sia parte attiva, anche per confermare il nostro rispetto e la nostra vicinanza ai nostri connazionali che, per ragioni di studio o lavoro, non hanno scelto, ma spesso sono stati costretti a lasciare il nostro Paese.

legge che, peraltro, questo Parlamento e il PD volevano cambiare - parole di Stefano Esposito, relatore del provvedimento sul codice degli appalti - togliendo il massimo ribasso al codice degli appalti, ma che - sempre per ammissione di Stefano Esposito - per interessi del PD, delle vostre Legacoop e delle vostre cooperative, avete ripristinato. Questo è il Paese in cui viviamo, al contrario: un Paese in cui il partito che doveva difendere i diritti dei lavoratori, li sfrutta, facendoci soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Li sfrutta rovinando i contratti, complici i sindacati, che continuano a firmare contratti da multiservizi da tre euro l'ora. CGIL, CISL e UIL, vergognatevi! Continuerò a denunciarlo, e voglio vedere a Torino, anche in campagna elettorale, se Fassino risolverà questo problema una volta per tutte. il sindaco di Bari, Antonio Decaro, pupillo del presidente Renzi e astro nascente del PD pugliese, sta dimostrando in questi giorni l'idea di sviluppo che questa maggioranza di Governo ha delle nostre città. Infatti, nella bellissima città di Bari, il caro Decaro ha deciso di fare abbattere 18 maestosi pini in via Caldarola, nel quartiere di Japigia, per far posto a magnifiche rotatorie in cemento, che costeranno ai poveri cittadini baresi ben un milione di euro: un esempio splendido dell'amore per il verde pubblico e per la salute dei cittadini. Altri venti alberi saranno abbattuti la settimana prossima. Ancora, nel progetto di rifacimento della rinomata via Sparano, sempre a Bari, il caro Decaro ha pronto un progetto che prevede l'abbattimento di ben 25 palme palme in favore di una inguardabile cementificazione pubblica. Insomma, i cittadini di Roma, Napoli, Torino e Milano sappiano quale modello di città ha in mente il caro Renzi, con i suoi fidi sindaci e candidati sindaci: meno verde e più cemento. A Bari il verde pubblico è già quasi inesistente. Tutti ne conoscono i benefici per la salute dei cittadini e la salubrità degli ambienti urbani, eppure il renziano caro Decaro, aspirante tagliaboschi, sperpera il denaro pubblico non per nuovi giardini dove far giocare i nostri bambini, ma per inutili opere in cemento, per aumentare la circolazione e l'inquinamento. Auguri a tutti!